di replica, innanzitutto per manifestare l'apprezzamento per il sensibile apporto che il Senato ha fornito al miglioramento di questo provvedimento, grazie grazie al paziente lavoro non solo del relatore, senatore Cucca, ma di tutta la Commissione, senza distinzione tra maggioranza ed opposizione. Anche il dibattito che c'è stato in Aula

che si occupa del complessivo riordino della magistratura onoraria, che è un pezzo importante del sistema giustizia, e pone fine al al sistema delle proroghe ripetute alle quali il Governo è stato costretto per superare l'emergenza. Durante il dibattito sono stati evidenziati alcuni elementi di criticità, che riguardano non tanto l'impianto generale del provvedimento quanto la disciplina transitoria. Alcuni di questi rilievi potranno essere superati con l'accoglimento da parte del Governo di alcuni degli emendamenti proposti.

«*Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente*: "*p)* ampliare nel settore penale la competenza dell'ufficio del giudice di pace ed ampliare nel settore civile la competenza del medesimo ufficio per materia e per valore, ed estendere per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500 i casi di decisione secondo equità"».

perché non c'è nessuna disciplina; non ci sono nemmeno i presupposti o i criteri perché possa individuarsi una disciplina.

il limite di 2.500 euro quando il magistrato giudica secondo equità. Ora, non è possibile andare a determinare un valore diverso da 2.500 euro, che non è più toccato nemmeno dagli emendamenti. Quindi, noi ci troveremo a scrivere un'affermazione che non è coerente con quanto viene votato successivamente.

e come si è già detto, è una norma di carattere generale che per l'appunto prevede l'ampliamento delle competenze del giudice di pace e, in relazione al contenuto della lettera *p)* esistente, lo aggancia al valore delle decisioni secondo equità. È tutto qua. Non si ravvisa assolutamente alcuna incongruenza rispetto al testo originario.

non è quello di opporci *sic et simpliciter* all'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia penale; di cercare di capire in ragione di quali criteri il legislatore delegato deve attuare questo tipo di ampliamento.

un minimo di criterio direttivo in ordine all'ampliamento della competenza penale del giudice di pace vi debba essere, altrimenti lasciamo completamente libero il legislatore delegato di ampliare a suo piacimento questa competenza, da cui poi - badate bene - scaturiscono delle condanne con possibili restrizioni in carcere se, per ipotesi, l'ampliamento è stato di carattere eccessivo. Nulla in contrario, a condizione però che vi sia un criterio direttivo.

chiedo scusa, cosa abbiamo votato? PRESIDENTE. Abbiamo votato prima l'emendamento 1.4, respinto, poi l'emendamento 1.5, respinto.

In questo senso, abbiamo fatto una proposta di sostituire l'ipotesi che non sia dovuto alcun tipo di indennità ai partecipanti al tirocinio con l'erogazione di una somma, che abbiamo variamente misurato nei vari emendamenti.

l'emendamento 2.105 che noi definiamo "evita esodati" relativamente al settore della magistratura onoraria. Tale emendamento si propone, al di là delle varie articolazioni delle tempistiche di rinnovo proposte nel disegno di legge, nei vari emendamenti del relatore e nelle ultime formulazioni, di assicurare a chi oggi è in carica, magari da molti anni, nei ruoli della magistratura onoraria e dei giudici di pace - e sappiamo quale sia l'importanza a livello a livello numerico e anche qualitativo dell'impatto sul contenzioso civile e penale del lavoro che svolgono i nostri magistrati onorari - la possibilità che fino all'età di settant'anni si possa provvedere al rinnovo

per le nuove assunzioni o discipline transitorie, si possa arrivare - com'è possibile - a casi in cui dopo lustri di onorato servizio non si raggiungano i requisiti minimi per maturare il diritto alla pensione con le casse

riteniamo che sia una formula di garanzia volta a sventare il rischio che si possano creare figure di esodati, cioè di chi magari dopo otto, dodici o più anni di servizio nei ruoli della magistratura onoraria si continuare a svolgere quell'attività, svolta ormai in maniera per lo più esclusiva, senza poter raggiungere i requisiti di età volti ad ottenere un trattamento pensionistico. Inoltre, Presidente, illustro

la magistratura onoraria. Sappiamo bene che si tratta di lavoratori sostanzialmente precari che non godono dei benefici di cui usufruiscono normalmente tutti gli altri lavoratori dipendenti, cioè non godono di maternità né di trattamenti retributivi a carico dello Stato perché

di facilitare coloro che opteranno per il servizio esclusivo alla magistratura onoraria, quindi rinunciando a svolgere o la libera professione di avvocato come spesso accade, o un eventuale

permettere di colmare i vari *vulnus* del trattamento lavorativo di cui soffrono i magistrati onorari. Nello specifico, si tratta di equiparare, disponendo un massimo di retribuzione,

questo servirebbe a compensare almeno parzialmente varie situazioni di sofferenza, che talvolta diventa anche di tipo esistenziale, ricordando che si tratta di lavoratori privi di tutte le tutele cui normalmente i lavoratori - almeno i pubblici dipendenti - godono. La qualifica, più precisamente, è quella di magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità, però, attenzione, senza possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria. È un beneficio, diciamo così, che noi vorremmo estendere a coloro che hanno almeno sei anni di anzianità di servizio. Insomma, dopo sei anni di magistratura onoraria, salvo procedimenti disciplinari o valutazioni sfavorevoli, il poter accedere a questo trattamento retributivo fino all'età di settant'anni, disponendo quel trattamento come un limite massimo, riteniamo che sarebbe certamente apprezzato dalle migliaia di giudici onorari, GOT, VPO e giudici di pace, che mantengono in piedi la macchina della giustizia. Ricordiamo che, stante la mancata possibilità o volontà da parte dello Stato o degli ultimi Governi, di provvedere a un piano di assunzioni, di riempimento dell'organico della magistratura togata,

sono le strutture che lo Stato concede loro, mantengono in piedi la baracca. Quindi, sarebbe dignitoso e meritorio un gesto, che il Parlamento volesse dare, di riconoscimento di diritti anche in questo caso.

Signora Presidente, vi chiedo un minimo di attenzione perché stiamo ragionando di una riforma che riguarda persone che danno un forte contributo all'amministrazione della giustizia, e lo fanno, molte volte, con sacrificio e senza essere neanche ben remunerati.

Il relatore dovrebbe informare che ha presentato degli emendamenti che modificano il primo periodo d'ingresso nella magistratura onoraria. Secondo quanto abbiamo votato in Commissione, il Governo, con un disegno di legge delega che molte volte fa acqua non avendo alcun criterio,

Il primo quadriennio viene diviso in due, per cui soltanto nel primo biennio è obbligatorio l'ufficio per il processo. magistrato onorario starà con un magistrato di carriera ordinario, che gli delegherà alcuni compiti mentre, negli altri periodi, svolgerà una funzione giudiziaria.

secondo la quale i Presidenti di quelle Regioni indicano le persone che devono essere nominate. Per questa ragione, con l'emendamento 2.24 propongo una regola particolare per quelle Regioni.

Per quanto riguarda l'ufficio per il processo, è evidente che va attivato per coloro che svolgono il primo periodo di attività, presentato l'emendamento 2.63. Siccome nella delega ci sono vari passaggi oscuri, bisogna chiarire che coloro che hanno maturato il primo quadriennio possono, in ragione di esigenze di servizio, essere ancora applicati per un periodo all'ufficio per il processo, periodo che, secondo oggettivi criteri di turnazione, non può però superare i sei mesi.

Ma non è scritto da nessuna parte come si determina l'indennità per coloro che svolgono l'attività giudiziaria. Quindi, non c'è nessun criterio.

poco) i vice procuratori onorari, i giudici onorari di tribunale e i giudici di pace.

a cui ho fatto riferimento. Nel 2013, dopo un lungo dibattito in quest'Aula, abbiamo eliminato la precedenza assoluta per chi svolgeva

che vadano a compensare le carenze riscontrate e ormai endemiche negli organici. E, nello stesso tempo, ci si vuole pilatescamente lavare le mani rispetto al futuro lavorativo dei soggetti

coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio, perché mi sembra veramente una dimostrazione di quanto poco sia rilevante ai fini della competenza, della partecipazione e anche dell'acquisizione di esperienza.

lo scenario futuro. Quando noi ipotizziamo due soli quadrienni o otto anni - come ha detto prima il senatore Caliendo - per chi fa una scelta proiettata nel futuro può avere un senso. Nell'emendamento 2.321,

che vale la fattispecie o il modello organizzativo che richiamava il primo il senatore Falanga per chi ha fatto il vice pretore onorario trent'anni fa perché, nel frattempo, la funzione è stata utilizzata diversamente. Ci sono stati rinnovi continui e, quindi,

Buccarella penso si pongano il problema di venire incontro alle legittime aspettative di chi deve essere accompagnato alla fine di un percorso lavorativo senza rete fino ad oggi - mi riferisco quanto meno a quella previdenziale e contributiva - che certamente non ha consentito alla stragrande maggioranza di questi operatori della giustizia di potersi arricchire, ma al massimo di poter dare un grande contributo in termini qualitativi e quantitativi, senza il quale l'attuale amministrazione della giustizia non può

magistrati onorari. Ritengo che questo criterio sia veramente molto aleatorio e generico e, quindi, gli emendamenti cercano di porre rimedio ancorando

associazioni dell'edilizia che chiedono di escludere dalle competenze dei giudici di pace quelle inerenti la materia condominiale, essendo

subordine all'esclusione delle materie condominiali dalla competenza di questi giudici, c'è la proposta di limitare l'importo, di mettere almeno un limite all'importo di queste cause, che sembra una soluzione più

del relatore, che incongruamente introduce nella delega l'istituzione di una forma di previdenza compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità.

di previdenza supplementare aggiuntiva e, per di più, irrigidendo questo tipo di di previdenza con delle norme di carattere generale. Non sentiamo davvero il bisogno di ulteriori norme, specialmente quando sono palesemente inutili, come in questo caso. Ecco perché proponiamo di sopprimere tale lettera dall'emendamento

prevedere che per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinarivigenti alla predetta data.».

vorrei ricordare all'Assemblea e ai signori senatori che in più di un'occasione questo problema è stato posto all'attenzione del Senato e in tutte le occasioni in cui questo problema è stato posto il voto del Senato è stato

senza alcun criterio di trasparenza al di fuori del voto di laurea, indipendentemente dall'università in cui quel voto di laurea è stato conseguito, abbiano sostanzialmente dei titoli preferenziali. Si era detto in passato che coloro che entrano nell'ufficio del processo possono fare direttamente il concorso in magistratura, senza essere avvocati, senza scuola di specializzazione, senza dottorato di ricerca e quant'altro e questa richiesta

rispetto agli altri vincitori di concorso; il che equivale sostanzialmente a prevedere la creazione di una strada assolutamente privilegiata nei confronti di soggetti che, come ho già detto prima, entrano senza criteri di trasparenza e che spesso, come diceva poc'anzi il senatore Caliendo, devono la loro entrata a rapporti di carattere amicale. Con questo emendamento il relatore dice che chi viene dall'ufficio del processo ha precedenza assoluta rispetto alle altre categorie, che pure hanno un certo tipo di precedenza. La domanda che vorrei rivolgere a voi se un soggetto che ha fatto parte dell'ufficio del processo è stato bocciato all'esame di avvocato, è stato bocciato al dottorato di ricerca, non ha conseguito il titolo di ricercatore universitario, è stato bocciato al concorso per notaio, sotto il profilo del merito è preferibile

prevedeva che una preferenza relativa nei confronti di questi soggetti, analogamente a chi ha il titolo di avvocato, di notaio o altro titolo può essere sufficiente. Non riesco davvero a comprendere la ragione per la quale questi soggetti debbano prevalere in modo assoluto rispetto ad altri che, attraverso il loro *curriculum* (già avvocati, già dottori di ricerca, già ricercatori universitari, già notai), hanno dimostrato, attraverso dei concorsi pubblici e, quindi, sostanzialmente attraverso criteri di trasparenza, di avere una preparazione assolutamente superiore a quelli che si sono limitati a fare l'ufficio del processo e, per ipotesi, sono stati bocciati all'esame di avvocato o di notaio, non hanno conseguito il dottorato di ricerca né il titolo di ricercatore universitario.

ad accantonare questo suo emendamento. Vede, signora Presidente, non so se il senatore Cucca sa quali siano le funzioni che svolge un giovane stagista all'interno dell'ufficio giudiziario. Credo che il senatore Cucca non lo sappia, proprio perché attribuisce un titolo preferenziale a costoro rispetto a un soggetto che svolge la professione da vent'anni.

fa uno *stage* nell'ufficio giudiziario, debba avere la precedenza su altri professionisti, che magari sono impegnati in attività professionale da anni. A me pare che, quantomeno, il senatore Cucca debba riflettere

È per questa ragione che, ove mai il senatore Cucca ritenesse di non ritirare l'emendamento 2.303 (testo 2), ritengo di potere dichiarare, a nome del mio Gruppo, che noi voteremo contro questo emendamento.

Questa era la realtà e oggi avremmo la stessa situazione. Abbiamo cercato di evitare che questa degenerazione proseguisse, introducendo una serie di concorsi con titoli e altri elementi, che si sono rivelati a loro volta farraginosi e comunque con delle pecche,

non si può definire precedenza assoluta, perché significherebbe veramente creare un canale privilegiato in cui - diciamocelo chiaramente - figli e parenti di magistrati ce li ritroveremmo magistrati onorari.

ha preso la mano perché nel tempo la magistratura onoraria è diventata sempre più necessaria. Poiché non veniva culturalmente ammesso

questa preferenza, che li mette in una posizione di privilegio, al di sopra di chi ha superato esami che gli hanno attribuito una professionalità riconosciuta dalle istituzioni dello Stato, a me sembra un'assurdità sul piano del sul piano del criterio dell'obiettività e della giustezza, incomprensibile agli occhi di chi frequenta ed ha conoscenza del mondo della giurisdizione e del diritto. Quindi, sul piano personale, annuncio il voto contrario su questo emendamento, per le ragioni che ho esposto. Signora Presidente, anch'io riprendo le considerazioni svolte dai colleghi fino adesso, a partire dal senatore Nitto Palma. Ricollegandomi a quanto diceva la senatrice Mussini, è vero che qui il criterio del merito è molto aleatorio e viene utilizzato come meglio conviene o come meglio crede il Governo, a seconda delle convenienze. Quanto diceva poc'anzi il senatore Torrisi penso sia da valorizzare e da tenere in considerazione. Io aggiungerei, senatore Torrisi, a quello che ha detto lei prima riguardo agli avvocati e ai

Ritengo che questo emendamento debba essere bocciato - e quindi annuncio il nostro voto contrario - proprio perché non c'è un concetto di merito univoco, ma viene utilizzato questo criterio

che un laureato in giurisprudenza, magari anche con i minimi termini, con una laurea presa molto alla leggera, debba giudicare un avvocato con un'esperienza di anni

perché un avvocato si deve trovare ad essere giudicato da qualcuno che non prenderebbe neanche come collaboratore gratuito nel proprio studio per fare le fotocopie? E arrivano continuamente emendamenti a tutelare il non

che va oltre la qualificazione dei migliori dei nostri talenti (invito i nostri colleghi a mantenere un giudizio cauto su questi talenti quando vanno all'estero), riteniamo

Nel suo intervento, il senatore Lumia ha asserito che il relatore, d'accordo con il Governo, ha presentato Senatore Lumia, il relatore, quando presenta un emendamento, non deve essere d'accordo con il Governo. L'accordo con il Governo non c'entra nulla e sarebbe, a mio avviso, anche un'attività scorretta quella di un relatore che, prima di presentare un emendamento, concordi

sarebbe sufficiente al fine di non creare problemi in relazione alle norme dello Statuto speciale che non solo prevedono la nomina da parte dei presidenti

che la soluzione che avevamo trovato in Commissione soddisfa l'esigenza a cui dovevamo mirare, e ritiro l'emendamento.

il merito delle questione. Nel merito non c'è alcun problema. Il testo dell'emendamento Caliendo è riproduttivo dell'attuale norma di attuazione. Mi riferisco alla legge n. 267 del 1992. Il punto è che non si può intervenire con una norma di rango ordinario per modificare o soltanto ripetere il contenuto di una disposizione di una norma di attuazione dello Statuto. È un problema di relazione tra fonti.

Presidente, prendo atto che il Governo e il relatore cambiano completamente prospettiva rispetto a tutto quello che è stato il dibattito di due anni.

parere. Probabilmente gli uffici del Ministero hanno deciso che bisognava tenere conto di ciò che rientrava nella mia proposta del 2011.

e lo trasformo in un ordine del giorno che, in sede di emanazione dei decreti attuativi, impegna il Governo a non determinare differenti indennità previste per le attività penali del giudice di pace sulla base dell'esito del procedimento. Chiedo cioè che il Governo, in sede di emanazione dei decreti attuativi, non preveda due diverse indennità, sia che il giudice di pace rinvii a giudizio l'imputato (l'indagato in quel momento) sia che adotti un provvedimento di proscioglimento.

Improvvisamente, quindi può capitare anche per ragioni di non accettazione di qualche decisione del giudice onorario, viene viene di nuovo spostato all'ufficio del processo, dove ritorna alle dipendenze e perde la titolarità della funzione giudiziaria. Non solo, egli regredisce a un'indennità più bassa

comportano eccezionalmente, secondo un criterio di turnazione, che si prendano i giudici onorari dei successivi bienni e si portino di nuovo a svolgere l'ufficio dei pregressi, almeno che questi non durino più di sei mesi. Vi è già un sacrificio, che sia almeno limitato nel tempo. Si vuol dire tre mesi? Ma lasciarlo così, alla discrezionalità più assoluta, credo che non sia un lavoro degno del Parlamento.

conto che vi sono persone che hanno dato molto in questi anni senza aver alcun riconoscimento per l'attività giudiziaria che si è potuta svolgere grazie al loro contributo. che ogni quattro anni saranno sottoposti a valutazione e che, quindi, devono essere confermati, salvo giudizio di demerito; pertanto non saranno confermati fino al settantesimo anno. Questa è la ragione per cui chiedo di sottoscrivere l'emendamento

Pertanto basterebbe andare a modificare la delibera dell'Ufficio di Presidenza che prevede questo e il problema sarebbe risolto: tenete pure le tessere dentro e nessuno verrà più a contestare la presenza della tessera. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È una cosa semplicissima e avremmo risolto il problema alla radice.

il tesserino inserito, ai fini amministrativi ha senso e significato nel momento della verifica del numero legale per il quale può esserci la presenza, ma la non partecipazione al voto che viene considerata ai fini amministrativi. la presenza del tesserino durante una votazione qualificata con il voto elettronico, ma in assenza dell'espressione del voto non produce alcun effetto amministrativo.

rischio di rimanere "esodati" nel momento in cui i rinnovi annuali o quadriennali ammissibili non potessero accompagnarli fino all'età pensionabile. A queste persone, che pure hanno sacrificato libere professioni o rapporti di pubblico impiego dai quali magari sono decaduti,

per svolgere quelle funzioni, mi domando perché per il giudice onorario debba prevedersi un'età diversa rispetto a quella dei togati.

la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative». Quasi a dire che essi devono fare un *part-time* di poco conto perché noi non possiamo pagarvi.

credo che anche chi non sia mai entrato in un palazzo di giustizia sappia che ai magistrati non si possono dare obiettivi.

prevedere che gli obiettivi di cui alle lettere *f)*, *g)* e *h)* devono essere individuate con riferimento al superamento della media di produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione Esiste un indice di produttività dei magistrati di un ufficio o di una sezione. Se si supera quell'indice, si avrà diritto alla parte variabile. Quindi non vi è una valutazione del singolo magistrato a cui si danno delle indicazioni e delle direttive che incidono sulla giurisdizione, ma gli si dice: alla fine dell'anno, se il tuo indice supera l'indice di produttività medio della sezione o dell'ufficio, hai diritto alla parte variabile. Guardate che è una cosa seria. Dire che si può valutare sulla base degli obiettivi significa ridurre la funzione giurisdizionale ad attività di amministrazione attiva.

vi prego di dare delle indicazioni su un aspetto che riguarda l'indipendenza dei giudici. Fate tante discussioni sulla Costituzione e sui principi di indipendenza, ma l'indipendenza - badate - non è solo del magistrato ordinario, ma anche del magistrato onorario. Per questa ragione vi chiedo di spiegarmi perché non può essere adottato un criterio che restituisca una dignità costituzionale al testo della delega.

Si è deciso che non sia opportuno fissare nella legge delega specifici criteri ai quali ancorare il riconoscimento della componente variabile dell'indennità, che l'emendamento da me presentato rimette

previste dal codice del processo amministrativo, in materia di incentivazione della produttività dei magistrati amministrativi, che rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi su proposta del presidente del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, previa delibera dello stesso consiglio, il compito di adottare, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure economiche

Il senatore Caliendo pone un problema importante: se non si specifica la natura degli obiettivi che vengono indicati al magistrato onorario, si corre il rischio che questi obiettivi possano in qualche modo attenere alla specifica attività del magistrato. Per cui io credo che l'emendamento del senatore Caliendo, che prevede l'inserimento rispetto al testo del relatore, possa anche essere riformulato nel senso di prevedere che gli obiettivi di cui alle lettere *f)*, *g)* ed *h)* non attengano alla specifica attività del magistrato onorario. secondo punto che voglio sottoporre all'attenzione del relatore è che, quando vengono posti degli obiettivi alla magistratura onoraria, il passo per porli alla magistratura ordinaria o alla magistratura amministrativa diventa estremamente semplice, con il forte rischio di andare ad incidere sull'autonomia e l'indipendenza della magistratura. XVII)*. Vedete, una cosa è dire che l'obiettivo è una riduzione del carico entro certi limiti accettabili; cosa diversa è invece porre un obiettivo che richiede, per essere raggiunto, un'attività di ufficio assolutamente insufficiente per il servizio che si deve rendere. Onde per cui io penso che, se il senatore Caliendo per ipotesi intendesse riformulare il suo emendamento, dicendo che gli obiettivi non riguardano la specifica attività del magistrato, il relatore sotto questo profilo

non potrà svolgere attività giurisdizionali, ovvero potrà farlo solo in taluni casi, su indicazione del giudice professionista. Così facendo,

alla disposizione che gli viene impartita dal giudice togato, che fine fa la sentenza? È valida, nulla o altro? Avete già previsto questo, che compromette in maniera seria l'autonomia e l'autonomia e l'indipendenza del giudice. Adesso il relatore, senatore Cucca, prende spunto da una disposizione che attribuisce

in via generale gli obiettivi che poi dà alla magistratura italiana.

avere anche degli obiettivi da raggiungere, che il senatore Caliendo, con l'emendamento presentato, cerca di fare in modo che non attengano alla specifica attività

dell'autonomia e indipendenza della magistratura. Se voi volete fare questo, sappiate che noi non intendiamo farlo e che vogliamo tutelare e proteggere i sacrosanti principi costituzionali dell'autonomia e indipendenza del giudice.

le affermazioni di chi, fino a poco tempo, fa ha fatto di tutto per imbavagliare e imbrigliare la giustizia mi sembra quasi ridicolo. Purtroppo - lo ribadisco - mi trovo nella situazione di dover condividere queste affermazioni, perché - purtroppo - ogni volta che si è ragionato sulla magistratura per obiettivi numerici, ne è venuto fuori un deterioramento degli obiettivi qualitativi e dei risultati. Sugli obiettivi qualitativi forse andrebbe fatto un approfondimento, cosa che difficilmente viene fatta negli ambiti previsti

vengono valutati solo sulla base di appartenenze politiche. Dove ci vorrebbe una valutazione effettiva non viene fatta e si va avanti per obiettivi numerici, dimenticando che l'attività del magistrato dovrebbe essere di altissima qualità,

per dare le progressioni in carriera in automatico a tutti i magistrati. Non ho mai visto un magistrato fermo al palo perché qualcuno gli ha detto che non era stato capace di fare il magistrato come si deve, cosa che invece sarebbe opportuno fare. Questo vale per la magistratura ordinaria e onoraria.

contiene un invito a sopprimere la lettera *i)*, che voglio leggere. Ogni volta che la leggo mi dico che non è possibile che si voglia fare una cosa del genere.

senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità. anni. Sono cose minime. È una sorta di assicurazione privata e c'è bisogno di una norma che dica che se noi troviamo un sistema ve lo consentiamo?

Vi prego, sopprimete la lettera *i)* perché un Parlamento non può arrivare a questi sotterfugi. O eravamo in condizione di risolvere il problema garantendo assistenza e previdenza o è meglio non scrivere nulla.

credo che con la parte dell'emendamento del relatore in cui si prevede di regolare «un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse mediante misure incidenti sull'indennità» si raggiunga il ridicolo.

evidentemente la possibilità che abbiamo avuto tutti noi delle opposizioni di formulare subemendamenti perfettamente articolati, anche dal punto di vista della copertura, va considerata con l'ovvia tolleranza della mancanza del tempo che ci è stato dato. Inoltre, rispondendo al senatore Cucca che non saprebbe come esprimersi su

Con il primo emendamento abbiamo detto che non si possono attribuire alla competenza dei giudici onorari le cause condominiali. Tutti voi conoscete la difficoltà delle cause condominiali e le diverse pronunce addirittura delle sezioni unite della Corte di cassazione.

nulla! Abbiamo la necessità di avere riforme che possano dare ai cittadini certezza dei propri diritti. Voi volete farlo, volete votare secondo ordini di scuderia: votate!

materia condominiale parte dalla validità della delibera condominiale che è un'operazione di analisi e di attenzione da parte del giudicante estremamente delicata, che attiene anche a profili di diritto amministrativo. Quindi, signori, la materia condominiale è particolarmente delicata ed ha ragione Caliendo quando dice che se guardiamo il repertorio noi troviamo impegnate le sezioni unite della Cassazione a decidere su questioni condominiali. Liberiamo i magistrati onorari da un compito, così difficile e faticoso, di decidere su cause di natura condominiale. Per questo noi votiamo a favore di questo emendamento.

siamo qui per parlare oltre che per votare.

Alcuni non hanno seguito nella precedente legislatura la riforma dell'ordinamento forense e non sanno cosa vivemmo. vorrei soltanto richiamare la vostra attenzione sul fatto che state votando una norma secondo la quale il magistrato onorario, che sarà confermato per quattro quadrienni quindi avrà acquisito una capacità e una preparazione per svolgere la funzione giurisdizionale superiore agli altri, per l'ultimo quadriennio dovrà ritornare a svolgere le sue funzioni esclusivamente

e solo eccezionalmente il Consiglio superiore della magistratura potrà autorizzarlo a svolgere le funzioni giurisdizionali. Rendetevi conto che state votando una cosa abnorme, fuori da qualsiasi logica. una persona che ha acquisito il massimo della professionalità dite: «Mettiti dietro». Credo che sia un qualcosa che non esiste tanto nelle aziende private quanto nella pubblica amministrazione. Poi venite a dire che volete fare

Caliendo ha posto l'accento sul profilo soggettivo dell'offesa che si rende a chi, dopo un lungo periodo di attività, nell'ultima fase: «Non devi svolgere più attività giurisdizionale, ma devi solo sopperire a quanto il giudice professionista dell'ufficio per il processo ti Ma io vedo la questione da altra angolazione. Non ritenete che noi abbiamo delle figure che alla fine non sono utili, non sono di aiuto nel raggiungere l'obiettivo che con la magistratura onoraria vogliamo raggiungere? Vi invito allora a riflettere bene. Sotto questi due diversi aspetti dovreste condividere l'emendamento del senatore Caliendo, se foste saggi. Noi lo siamo e lo condividiamo.

sull'esercizio dell'attività dei magistrati per una loro conferma e nomina. Di questo stiamo parlando? Quindi il Consiglio giudiziario, che ha una sua sezione apposita ed autonoma in cui sono già rappresentati i giudici onorari, l'ordine degli avvocati e i professori universitari,

Signor Presidente, senatrici e senatori, ieri in Svizzera chiudeva gli occhi per sempre la signora Susanna Zambruno Martignetti, una donna forte che ha lottato contro la sclerosi multipla per venticinque anni. La signora Susanna ha deciso di porre fine alla sua vita e alle sue sofferenze in modo volontario e per farlo ha dovuto abbandonare il suo Paese, l'Italia, per andare in Svizzera. Originaria di Torino, lascia un figlio di venticinque anni, un marito che le è stato sempre accanto e una sorella che ha voluto essere presente in ogni istante. Loro, pur non condividendo il desiderio della signora Susanna, l'hanno comunque assecondata. La sua scomparsa getta un'ombra sulla legislazione italiana, che ancora non permette ai cittadini di lasciare i propri cari con dignità e coraggio, perché un gran coraggio è servito a Susanna per compiere questo gesto, lontano dalla sua casa e dalla sua città. L'eutanasia non è una parola che deve far paura, ma una scelta compiuta in piena coscienza quando dolore e sofferenza hanno ormai il sopravvento e mascherano le gioie della vita. Il 1° marzo alla Camera dei deputati sono stati assegnati due disegni di legge alle Commissioni 2ª e 12ª riunite, che fanno riferimento alla proposta già sostenuta dai cittadini nel 2013 per la legalizzazione di procedure che trovo indispensabili in una società aperta di vedute. Nostro compito, infatti, è tutelare e rispettare le volontà di coloro che scelgono una morte dignitosa, senza accanimenti terapeutici. L'Italia necessita di una legge che regolamenti almeno il fine vita e, più coraggiosamente, anche l'eutanasia e che permetta a persone come Susanna Zambruno Martignetti di morire a casa propria, circondata dagli affetti e da un ambiente familiare. Sottolineo che si tratta anche di un problema di equità, perché chi ha condizioni economiche personali e familiari che lo consentono può permettersi di andare in Svizzera e spendere oltre 10.000 euro, mentre chi non può permetterselo, come al solito non può decidere del proprio destino. Dobbiamo riconoscere i limiti della medicina e concludo chiedendo a tutti quali siano le motivazioni che impediscono questo importante passo per la nostra legislazione. Rispetto profondamente tutti coloro che pensano che non ricorreranno mai a questa possibilità né per sé, né per i propri familiari, ma chiedo lo stesso rispetto verso chi vuole fare una scelta diversa, a cui viene impedita. Credo che, mettendoci nei panni di chi soffre, occorra affrontare con coraggio il tema dell'eutanasia per far sì che persone come Susanna non siano più costrette a recarsi all'estero per porre fine alla propria vita, vita, senza considerare - lo ripeto - che una legge sarebbe una misura equa nei confronti di chi non ha possibilità economiche di andare in Svizzera.

per informare tutti voi della situazione che stanno vivendo ancora una volta i lavoratori della ex Indesit-Whirlpool. Ci spiace infrangere la favoletta raccontata dalla Whirpool attraverso frequenti comunicati stampa per dirvi che la situazione è ben diversa da come viene descritta. L'azienda, infatti, avendo ricevuto con gli ultimi accordi una serie di agevolazioni e facilitazioni milionarie, ora ha la necessità di mostrare che tutto va bene e scorre per il verso giusto. Ne saremmo lieti se ciò corrispondesse al vero, ma così non è, perché noi del Movimento 5 Stelle facciamo una cosa che questo Governo non ha mai fatto: ascoltare i lavoratori che ci raccontano di una situazione sempre più insostenibile nel Casertano, ma non escludiamo - anzi abbiamo forte preoccupazione che la situazione sia identica anche negli altri stabilimenti ex Indesit. Abbiamo deciso, quindi, di depositare un'interrogazione per avere maggiori informazioni da parte di quei soggetti istituzionali che sono stati e sono coinvolti direttamente nell'attuazione degli accordi e del piano industriale. È noto a tutti che questo Governo è esperto nel fare promesse per poi disattenderle, soprattutto quando si tratti di diritti dei cittadini e dei lavoratori e non di potenti *lobby* o banche. Per vari mesi abbiamo denunciato, anche in questa Aula, il mancato rispetto dell'accordo del 2013. Ebbene, ora dobbiamo constatare che neanche stavolta si stanno rispettando gli impegni presi con l'accordo siglato a luglio 2015. Ad oggi non ci risultano infatti realizzati gli investimenti, né i trasferimenti, né i prepensionamenti; non sono stati attivati appositi non sono iniziati i lavori di riconversione dello stabilimento di Carinaro; né cedute o affittate le aree, i terreni e gli *asset* di proprietà a condizioni vantaggiose; né sono stati attivati programmi di riqualificazione del personale. Infine, Presidente, per noi l'accordo quadro formalizzato il 24 luglio 2015 risulterebbe in gran parte disatteso e non comprendiamo quale sia il futuro degli oltre 800 lavoratori di Carinaro, quanti siano gli esuberi, i prepensionamenti, i trasferimenti e quali i costi sostenuti dallo Stato italiano. italiano. Forse - e dico forse - sarebbe opportuno che anche il Governo si preoccupasse dei lavoratori italiani così come da sempre fa il Movimento 5 Stelle.

come quelli che sono stati sollevati a fine seduta (l'eutanasia, il fine vita, le cure palliative, l'accanimento terapeutico) non possano essere sviluppati nell'Aula del Senato partendo da un caso specifico

fissando anche limiti e ambiti delle cose di cui stiamo discutendo, che non riguardano una sola persona, ma fenomeni come, per esempio, quelli del Belgio, dove c'è una moltiplicazione esponenziale di coloro che

condivisa tra tutte le forze politiche, senza anticipare conclusioni che devono invece essere approfondite in un dibattito, vista la delicatezza della questione. Presidente, spero che ci siano i luoghi adatti, in Commissione e in Assemblea, alla Camera e al Senato, per approfondire queste tematiche che sono assolutamente delicate e richiedono un approfondimento. Signor Presidente, colleghi, pongo una questione importante. Da alcune settimane è in corso in molti atenei italiani una campagna di mobilitazione del Coordinamento nazionale ricercatori e ricercatrici non strutturati per il riconoscimento della ricerca come lavoro. L'iniziativa, denominata «Sciopero alla rovescia», nasce in seguito alla bocciatura da parte della Commissione bilancio della Camera dell'emendamento per l'estensione dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) ai ricercatori e alle ricercatrici precarie. Peccato, perché questa era una promessa che il Governo aveva fatto e su cui aveva espresso anche parere favorevole, ma poi se l'è rimangiata. Con questa decisione, infatti, il Governo, contrariamente a quanto sancito dalla Carta europea dei ricercatori, si è rifiutato di estendere il diritto a ricevere l'indennità di disoccupazione prevista per gli altri lavoratori parasubordinati. Stiamo parlando di un diritto acquisito che dovrebbero avere. Per rispondere a questa ennesima delegittimazione del lavoro accademico, negli ultimi giorni, dal 2 febbraio, è stato lanciato uno "sciopero alla rovescia", ovvero uno sciopero bianco, durante il quale i ricercatori e le ricercatrici non strutturati indossano la maglietta rossa,

borsisti e dottorandi, a fronte di 50.000 strutturati - quindi più della metà degli impiegati all'università - che tengono lezione, organizzano convegni, fanno ricerca, mandano avanti i laboratori e propongono progetti internazionali con successo. Cosa chiedono?

attualmente pari appena allo 0,5 per cento del PIL nazionale, ovvero meno della metà della media dei Paesi europei: complimenti! Sono fondamentali lo sblocco del *turnover* e un piano di reclutamento straordinario. Dal 2008 sono stati 10.000 i pensionamenti di docenti strutturati e c'è stato il blocco del *turnover* e nei prossimi cinque anni ne spariranno altri È evidente che è in atto un sistema per chiudere gli atenei e distruggere l'università pubblica. È, quindi, necessario rispondere con determinazione alla volontà di una parte politica di smantellare il carattere pubblico dell'università: o stabilizziamo questi lavoratori e investiamo nella ricerca, oppure è questione di mesi e l'università pubblica e la ricerca moriranno. Ma forse è questo il progetto di Renzi. Signor Presidente, ho appena presentato un'interrogazione parlamentare sull'inquietante vicenda di Seregno, un Comune vicino al mio, in Brianza. Il prefetto ha chiuso due bar, perché i proprietari risultano in contiguità con la 'ndrangheta e alcuni sventurati hanno appeso un lenzuolo di solidarietà, con le immagini non delle vittime di mafia e 'ndrangheta, ma dei proprietari del bar. Seregno, ci sarà una manifestazione contro le mafie, cui do il mio convinto incoraggiamento, tanto più che mi risulta che la polizia giudiziaria, l'altro giorno, ha svolto un'acquisizione documentale presso il Comune di Seregno e l'ufficio del sindaco Mazza. Per questo Per questo sono ansiosa di conoscere la risposta del Governo alla mia interrogazione. Signor Presidente, colleghi, nell'agenda del Governo dovrebbe rientrare, fra le priorità, la delicata e preoccupante questione legata a Finmeccanica in Puglia e a tutto il comparto aerospaziale della Regione, del quale - ci tengo a precisarlo - fanno parte numerose piccole e medie aziende, che rappresentano il tessuto economico della mia Regione. Vorrei sollecitare, attraverso questa nota, l'avvio di un'indagine conoscitiva, sottoposta dal sottoscritto alla Commissione industria del Senato. Soprattutto alla luce dei fatti degli ultimi giorni e dopo gli esiti dell'ultima riunione tenutasi in Confindustria a Brindisi, fra Finmeccanica Divisione elicotteri e le varie sigle sindacali, appare indispensabile e urgente un intervento conoscitivo. Non possiamo perdere ulteriormente tempo: occorre convocare, con estrema urgenza e prima che diventi troppo tardi, i vertici del colosso industriale e delle altre aziende del settore. I continui scioperi dei lavoratori delle aziende del distretto e il numero crescente dei lavoratori senza prospettive future ci impegnano a verificare il piano industriale di Finmeccanica. Le logiche industriali e di mercato messe in atto stanno portando al collasso l'intero comparto aerospaziale pugliese, considerato da sempre uno dei settori strategici per tutta l'economia territoriale. La volontà di delocalizzare, che di fatto vuol dire trasferire degli interi settori all'estero, chiudendoli in Italia, sta mettendo a rischio la tenuta di tutte quelle piccole e medie imprese che si interfacciavano con il gruppo di Finmeccanica e sta mandando a casa centinaia di lavoratori, che da oggi non avranno più un'occupazione e si vedranno privati del loro lavoro e della loro professionalità. Dovremo chiederci il perché di queste scelte, perché Finmeccanica vuole chiudere in Italia e delocalizzare in Polonia. Il Governo, l'Italia, i cittadini e quei lavoratori devono conoscere le motivazioni di questa decisione. Le ripercussioni sul tema del mercato e sul livello occupazionale di tutte quelle realtà ci impongono di fare una vera riflessione sulla politica che Finmeccanica attua in questa materia. È a rischio il futuro di centinaia di lavoratori e di famiglie.

che investe solamente un terzo della somma totale con fondi propri e rimane proprietaria dell'infrastruttura. Sono in corso delle indagini della magistratura relativamente ad alcuni dipendenti, sollecitate

avere delle informazioni, visto che il Governo ha stanziato 2,2 miliardi di euro per fare l'infrastruttura in questione e dice di volerla realizzare attraverso Infratel.

per tutelare i cittadini e i soldi pubblici, che non devono finire nelle tasche di un privato, che rimane sempre e comunque dominante sul mercato. Vogliamo fare queste cose? Bene, il Governo risponda all'interrogazione e ci attendiamo che agisca con vigore, se ne è capace.